Grazie,

Grazie,

Signor Presidente, colleghi, le Commissioni bilancio e sanità non hanno terminato l'esame degli emendamenti e non hanno quindi conferito il mandato ai relatori per riferire in Aula. A questo esito si è giunti, da un lato e principalmente, per la legittima attività ostruzionistica di una parte delle opposizioni e, dall'altro lato, per gli effetti della prassi che vuole che le Commissioni non si riuniscano nei giorni in cui non si tengono impegnative sedute d'Assemblea. Quanto al primo punto, l'ostruzionismo, sarà la discussione generale a chiarirne le motivazioni e a consentire a tutti, qui dentro e fuori, la formulazione di un giudizio. A me compete solo mettere in evidenza che esso si è sviluppato nel rigoroso rispetto del Regolamento e che il presidente Marino ed io abbiamo preso atto della impossibilità di concludere i lavori solo ore 23,10 di ieri, quando cioè il computo matematico dei tempi di esame e votazione degli emendamenti che rimanevano da esaminare ha mostrato che sarebbero state necessarie ulteriori 24 ore di lavoro; 24 ore che non erano nelle nostre disponibilità perché appunto questa mattina sarebbe cominciata la relativa seduta.

l'esperienza di queste settimane ‑ se ce ne fosse stato ancora bisogno ‑ non fa che confermare l'urgenza dell'applicazione di quanto previsto dall'ordine del giorno presentato dai Presidenti delle Commissioni ed approvato proprio in occasione della discussione sul bilancio del Senato. Lei ricorderà, signor Presidente, che in quella occasione tutti i Presidenti delle Commissioni permanenti hanno sottolineato l'esigenza di organizzare i lavori delle Commissioni secondo calendari che non si limitino ad occupare a questo scopo la parte residua e gli interstizi dei lavori dell'Aula, sospendendosi nelle nelle settimane in cui l'Assemblea effettivamente non affronta riunioni e decisioni impegnative. Se si applica questo schema, qualsiasi qualsiasi attività ostruzionistica, anche la più lieve e organizzata senza particolare intensità, è in grado di impedire alle Commissioni di sviluppare il loro lavoro. Ma più in generale, al di là dell'ostruzionismo, ciò che viene in evidenza è che il lavoro delle Commissioni risulta troppo compresso. Abbiamo approvato, in sede di discussione del bilancio del Senato, un ordine del giorno in questo senso.

che hanno accumulato disavanzi nel periodo 2002-2005. La discriminazione è fondata sul fatto che solo alcune Regioni, quelle più inefficienti e meno capaci,

è manifestamente irragionevole il criterio selettivo utilizzato per regolare l'accesso delle Regioni in disavanzo). Si viola poi il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo in quanto pubblici uffici, sono chiamate costituzionalmente ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione. Tale obbligo assume un peculiare rilievo nel settore sanitario che, come noto, impiega l'80 per cento dei bilanci regionali. Il provvedimento, finalizzato a sanare l'inefficienza cronica di alcune Regioni, rappresenta un'evidente negazione del principio costituzionale disincentivando le Regioni cosiddette

riservando allo Stato una competenza esclusiva alla sola determinazione dei livelli essenziali di assistenza. Anticipando tale riparto costituzionale l'articolo 8 del decreto legislativo n. 56 del 2000, sopprimendo il tradizionale Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata, ha eliminato nei confronti delle Regioni il previgente vincolo di destinazione. Nel nuovo assetto costituzionale si ritiene conseguentemente preclusa per lo Stato la possibilità di attribuire alle Regioni in materia di potestà concorrente finanziamenti a destinazione vincolata, come i 3 miliardi oggetto di riparto nel decreto-legge in titolo. Segnalo poi la violazione del principio dell'autonomia e responsabilità finanziaria regionale, di cui all'articolo 119 della Costituzione: lo straordinario intervento statale si pone palesemente in contrasto con i princìpi sull'autonomia e la responsabilità finanziaria di ciascuna Regione. In particolare, il quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione prevede la possibilità che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali a favore di determinate Regioni solo «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali». violazione del principio di leale collaborazione, di cui all'articolo 120 della Costituzione: è evidente che il principio di leale collaborazione tra gli enti territoriali ha portato a un nuovo spirito cooperativo incentrato sulla stipula periodica

disperati perché dovevano pagare qualche corso per veline e qualche viaggio all'estero in prima classe a spese dei contribuenti. Allora, magari, il criterio d'urgenza forse

per il semplice fatto che, storicamente, abbiamo Regioni povere e Regioni ricche. Sgombriamo il campo da queste falsità. Oggi in Italia le Regioni ricevono all'inizio, euro più euro meno, la stessa quota *pro capite*, cioè gli stessi soldi per ogni cittadino che deve essere assistito dal punto di vista sanitario. Quella che cambia successivamente è la capacità di utilizzare questi soldi e, quindi, l'efficienza dei vari sistemi sanitari regionali; tant'è vero che la Lombardia, che a detta di vari istituti di certificazione stranieri certamente la migliore sanità pubblica, insieme a qualche altra Regione italiana, e una delle migliori sanità europee, sempre nel campo pubblico, alla fine chiude i propri bilanci in pareggio, nonostante ciò che qualche Ministro dichiara in televisione. Per realizzare tale pareggio di bilancio non ha a disposizione più risorse della Regione Campania o della Regione Lazio, perché si tratta di 1.400 euro all'anno circa per ogni lombardo,

di crediti nei confronti di altre Regioni, che ormai sono diventati sostanzialmente inesigibili. Detto ciò, la differenza sta nell'efficienza dell'utilizzo del denaro. del denaro. Non intendo farne una questione di destra o di sinistra, di chi c'è stato prima o di chi ci sarà dopo perché oggi parliamo di debiti dal 2000 al 2005, però dal 2005 al 2007 i dati provvisori dicono che nella Regione Lazio il disavanzo continua ad andare avanti esattamente come prima. Intendo parlare semplicemente della capacità del sistema socio-economico di ogni Regione di far funzionare o meno il proprio sistema sanitario. Ebbene, a fronte di tale situazione che porta, ad esempio, una Regione come la Lombardia ad essere in perfetto pareggio, abbiamo altre Regioni che invece perdono 3, 4, 5, 10 miliardi di arretrati, come la Regione Lazio. Con questo provvedimento non si individuano le cause di questa differenza di efficienza tra una Regione e l'altra. Si mette semplicemente una pezza e con voi è la terza pezza che in pochi mesi mettiamo al sistema sanitario, come se continuando a mettere pezze i problemi si risolvessero da soli. La Regione Lazio ha accumulato 10 miliardi di debiti negli anni precedenti, che andremo a coprire con 2 miliardi adesso e con altri 6 miliardi che lo Stato graziosamente presta con una restituzione presunta forse in trent'anni (quindi con un mutuo mascherato che la Cassa depositi e prestiti fortunatamente almeno non ha voluto concedere per carità di patria, oltre che per un minimo buonsenso). Diamo un miliardo alla Regione Campania; però nel frattempo la Regione Lazio sta continuando ad accumulare ogni anno esattamente gli stessi debiti che hanno portato sul bilancio corrente ad avere oggi 10 miliardi di debito complessivo. Quindi eroghiamo a fondo perduto delle diamo un prestito di 6 miliardi ulteriori che dovrà essere restituito in parte ogni anno per trent'anni, ma nel frattempo ogni anno continuiamo ad accumulare debiti. Come facciamo ad uscire da questa situazione se nel provvedimento non c'è il minimo richiamo al senso di responsabilità di chi gestisce?

un minimo di buonsenso costituzionale. L'unità d'Italia quando fa comodo la si sventola in tutte le salse, mentre quando non fa comodo la si dimentica. Perché i lombardi devono pagare il *ticket* e i laziali no?

Regioni dove si pagano le tasse e Regioni dove non si pagano le tasse. L'IRAP, che dovrebbe essere una tassa nazionale che serve a coprire in gran parte la spesa sanitaria, la si paga per l'85 per cento sotto il Po l'IRAP non esiste. L'IRAP - ricordo - come minimo è il 5 per cento del monte salari e il monte salari e stipendi c'è in tutta Italia. Siccome i disoccupati

nessuno dice. Per non parlare, visto che voi siete federalisti, del Fondo di solidarietà nazionale in materia sanitaria, ossia altri 6-7 miliardi che vanno sempre nel calderone, che si aggiungono ai 1.400 euro a testa di cui si diceva all'inizio. Qualcuno qui mi deve spiegare, soprattutto i sostenitori del Tricolore e dell'Unità d'Italia, perché i lombardi, che alla fine sono dei poveracci che lavorano dalla mattina alla sera, devono pagare il 57 per cento di questo fondo nazionale. Ditemi come fa ad essere nazionale un fondo che è pagato al 57 per cento da un'unica Regione, mentre tutto il resto viene pagato da altre tre o quattro Regioni; però, si distribuisce gratis a tutte le altre.

che non è capace di tirar su i sacchetti della spazzatura per strada, che dice che ha firmato i contratti ma non li aveva letti perché non aveva tempo, che fa i concorsi per veline o spende non so quanti milioni di euro

Chi spende paga, il fondo di solidarietà serve per le emergenze, serve per ciò che oggettivamente le Regioni più povere non possono coprire, non per pagare gli sprechi che chi non è chiamato a rispondere si permette di continuare a fare. Riteniamo che non vi sia alcuna urgenza, a fare. Riteniamo che non vi sia alcuna urgenza, perché comunque stiamo parlando di una questione di anni fa. Con qualche settimana in più di discussione in Commissione (smettendola con la consuetudine di far arrivare i provvedimenti al Senato quando mancano poche ore alla loro scadenza, per cui non si ha mai tempo

Presidente, onorevoli colleghi, da anni il Gruppo della Lega Nord si batte per decentralizzare competenze su attività relative alla fornitura di servizi e di prestazioni pubbliche, così da tenere così da tenere adeguatamente conto delle specificità locali. In materia socio-sanitaria la legislazione ordinaria vigente consente alla Regioni di sviluppare un sistema di assistenza sociale e di tutela della salute che segue da vicino le esigenze della collettività locale. In particolare, il decreto legislativo n. 56 del 2000 ha segnato un passaggio fondamentale nell'autonomia fiscale delle Regioni sopprimendo i fondi vincolati statali ed attribuendo alle Regioni «risorse locali» a copertura delle spese sanitarie IRAP, IRPEF, e le risorse stornate da altri capitoli del bilancio regionale): da allora il debito ricade sotto la responsabilità e la capacità di gestione delle Regioni stesse. In tale ottica il decreto-legge oggi in esame non può che suscitare parecchie perplessità. Il nuovo intervento di ripiano finisce per far pagare per la terza volta allo Stato i disavanzi sanitari regionali: si ricorda che un primo intervento era stato disposto dalla finanziaria 2006, che aveva stanziato 2.000 milioni di euro per il 2006 per la copertura dei disavanzi pregressi del Servizio sanitario

subordinatamente alla stipula di un'intesa Stato-Regioni per il contenimento delle liste di attesa; a questo intervento si aggiunge il Fondo transitorio istituito dalla legge finanziaria 2007, Presidente, sono costretto a difendere la dignità e la libertà dei miei senatori ad intervenire

e/o nelle quali sia scattata l'applicazione ai massimi livelli delle addizionali ed aliquote regionali. Ne consegue un'evidente sovrapposizione di operazioni statali di ripiano, destinate indubbiamente a scoraggiare l'effettivo risanamento dei conti regionali e ad indebolire anche le aspettative delle Regioni «virtuose» circa la serietà del patto stipulato con lo Stato. Inoltre, i criteri del ripiano di 2,3 miliardi di debiti della sanità, proposto dall'attuale Governo di centro-sinistra, riducono di fatto solo a quattro le Regioni che possono accedervi. Nello specifico si tratta della Regione Lazio, che negli ultimi tre anni aveva accumulato un *deficit* di 3,9 miliardi di euro, della Campania, dell'Abruzzo, e della Liguria. A prescindere da come la si voglia presentare, quest'ennesima operazione di assistenza nazionale alle «deboli» Regioni del Sud e al Lazio, contiene un'unica lettura possibile: ancora una volta il Governo ricompensa l'irresponsabilità gestionale di poche Regioni che, a differenza delle altre, non si sono mai mosse con iniziative proprie e continueranno a non farlo, finché possono fare sempre affidamento sulla benevolenza dello Stato. Che non si tratti di pregiudizi lo dimostra ampiamente uno studio, condotto dalla Cergas-Bocconi e pubblicato lo scorso novembre, in cui si attesta che il disavanzo sanitario nazionale è determinato sempre dalle stesse Regioni, cioè quelle che accettano l'affiancamento ministeriale. Peraltro, tali Regioni, secondo le più recenti stime sull'ammontare dei disavanzi sanitari regionali, non solo non hanno risolto, ma registrano un continuo peggioramento nei saldi di bilancio, al contrario delle numerose altre Regioni che, pur avendo accumulato disavanzi tra il 2002 e il 2005, hanno provveduto autonomamente a coprire tale situazione di *deficit*. Le Regioni hanno tre strumenti principali per il controllo della spesa sanitaria: l'aumento delle entrate tributarie, attraverso i *ticket*, la maggiorazione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF e, infine, le risorse stornate da altri capitoli del bilancio regionale. Possono operare, dunque, dal lato della spesa, delle entrate fiscali o di entrambi, oppure possono lasciar lievitare il *deficit* contando sull'assistenzialismo. È senz'altro il caso del Lazio, che, dopo le elezioni del 2005, con la nuova giunta di centro-sinistra, pur presentando percentualmente la più elevata spesa farmaceutica, ha eliminato il *ticket* all'assistenza farmaceutica similmente all'Abruzzo. Il risultato di queste scelte puramente ideologico-demagogiche è che tra il 2003 e il 2005, il Servizio sanitario nazionale ha accumulato quasi 13 miliardi di disavanzo,

Osservando l'andamento delle Regioni nel triennio 2003-2005 esiste però, tra esse, anche un gruppo che, contando solo sulla propria capacità di controllo della spesa, senza ricorrere all'imposizione fiscale, è riuscito a contenere il *deficit* su bassi livelli. (Lombardia e Veneto), poi, puntando sul controllo della spesa sanitaria e ricorrendo, in aggiunta, all'imposizione fiscale, oppure a risorse autonome di bilancio, hanno disavanzi minimi o addirittura degli avanzi. A quanto pare, una gestione responsabile delle proprie risorse ed un valido controllo della spesa permettono, dunque, di incidere sensibilmente sul *deficit* sanitario. È perciò doveroso che oggi questo Governo ponga fine ad un sistema sbagliato che ricorre da troppo tempo, ovvero che in questo Paese il rigore non è premiato. Non è possibile continuare in un atteggiamento assistenzialista che, oltre ad essere diseducativo ed ingiusto per i contribuenti, ha rivelato, a più riprese, la sua inefficacia. L'emblematico caso del Lazio pone in evidenza l'urgenza che gli elettori compiano una scelta responsabile ed oculata al momento del voto dei propri governanti, ma anche che vengano sanzionati soprattutto gli amministratori e i politici che non hanno saputo o voluto compiere scelte responsabili per il mantenimento in attivo del proprio sistema sanitario. È necessario promuovere la responsabilità dei comportamenti: le Regioni del Nord non possono continuare a sostenere le proprie spese, mentre quelle del Centro e del Sud non tentano nemmeno di impegnarsi nel controllo della spesa. È troppo facile assicurarsi il consenso il consenso a spese di quelle Regioni che, pur avendo prodotto un disavanzo, si sono immediatamente e responsabilmente premurate di coprirlo attraverso un innalzamento della pressione fiscale (Piemonte, Veneto). È ora che lo Stato intervenga contro chi, per incapacità o inadeguatezza, ha generato o aggravato una situazione di *deficit,* imponendogli di rinunciare alla propria carica. Questo sarebbe un segnale importante ai fini di un riconoscimento meritocratico, non solo nei confronti degli amministratori regionali, ma anche dei cittadini che li hanno eletti. Al contrario, il decreto-legge oggi in esame si pone in continuità con un'ottica assistenzialista e antifederalista. *(Applausi

colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, inizio subito con questo dato: gli italiani che possono non si fanno curare in Italia. Preferiscono andare altrove, persino nella Repubblica Ceca. Del resto, significherà qualcosa che il 64 per cento degli italiani ritiene che la riforma del Sistema sanitario nazionale sia non solo necessaria, ma anche urgente; cento si dichiari insoddisfatto della qualità delle prestazioni sanitarie e che il 71 per cento pensi che la situazione tra dieci anni sarà addirittura peggiore. Solo il 18 per cento degli italiani giudica accettabili i tempi di attesa per esami e visite specialistiche, mentre appena il 30 per cento ritiene sufficiente l'informazione riguardo temi inerenti salute e cure sanitarie. Questi sono dati recenti, del febbraio di quest'anno, che emergono da una recente indagine internazionale che ha esaminato, oltre all'Italia, la Francia, la Spagna, l'Olanda, la Germania, la Gran Bretagna, la Repubblica Ceca e la Svezia. Questa inchiesta ci offre l'immagine di un Paese, il nostro, non solo assai deluso dal proprio sistema sanitario, ma anche scettico e prevenuto quando si parla di ospedali e *ticket* sanitari. Di fronte alle differenti ipotesi di riforma, è interessante rilevare come i molti problemi del Sistema sanitario nazionale inducano una larga parte degli italiani (quasi il 70 per cento) ad esigere un più stretto controllo sulla spesa pubblica, ma un numero non molto inferiore (oltre il 50 a chiedere la possibilità di destinare più risorse private nella spesa sanitaria e a pretendere (oltre il 60 per cento) una maggiore libertà di scelta del medico e degli ospedali. Malgrado questi dati - una generale sfiducia nella gestione pubblica della sanità e un alto tasso di fughe all'estero per farsi curare gli italiani, nella maggioranza dei casi, restano attaccati all'idea dello Stato sociale e al principio di uguaglianza rispetto alla salute. Non è facile spiegare che l'universalità delle prestazioni deve essere garantita solo dallo Stato, il quale, peraltro, non è più in grado di soddisfare le esigenze degli utenti. Non solo, sarà anche necessario introdurre criteri di competitività tra centri di assistenza, stilando vere e proprie classifiche sulla qualità delle prestazioni che stimolino a migliorare l'offerta e diano indicazioni agli utenti, anche per orientare le loro libere scelte. Insomma, cari colleghi, per uscire dall'inflazione sanitaria e migliorare la qualità dell'assistenza medica, la strada da percorrere è quella del mercato e della competizione e non dello smantellamento della sanità privata che spesso riesce a recuperare quelle sacche di stagnazione che il sistema pubblico spesso in questo ultimo anno ha generato. Senza un cambiamento preciso la sanità in Italia va incontro al disastro, come quello che ha vissuto l'Inghilterra nel 2002. Dobbiamo dunque imparare dalle esperienze degli altri, in particolare dall'esperienza inglese, altrimenti anche noi commetteremo lo stesso errore. Nel 1948 l'Inghilterra aveva creato un sistema assolutamente interessante, ma che negli anni non ha saputo modificarsi, a tal punto da essere schiacciato dal dissenso stesso dei suoi cittadini.

Questo ci impegna ad essere flessibili e capire che il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare per essere all'altezza dei tempi. Il nostro Paese ha intrapreso un percorso culturale, prima che pratico e organizzativo: una grande opportunità per migliorare la nostra sanità e i servizi offerti al cittadino. Ma solo un personale aggiornato può erogare prestazioni di qualità e contenere l'uso inappropriato delle risorse. Questo Governo ha addirittura tagliato gli ECM. È inaudito! Nonostante Nonostante norme e direttive sanitarie, anche recenti, che imponevano una drastica diminuzione dei tempi d'attesa per esami diagnostici ed operazioni chirurgiche nell'ambito della sanità pubblica, la realtà è purtroppo ben diversa. I risultati della IX Relazione del Piano salute di «Cittadinanzattiva» non sono certo esaltanti: il dato più inquietante riguarda proprio i tempi d'attesa. Pensate, colleghi: per un intervento chirurgico oncologico si arriva fino a 120 giorni di attesa. Chi non vuole o non può aspettare deve rivolgersi alla sanità privata, ma non tutti hanno disponibilità sufficiente di denaro e sono per questo costretti ad indebitarsi. Un'altra nota dolente riguarda i farmaci di classe C, classe famosa perché sono i farmaci che dobbiamo pagare, di cui si è molto discusso, e che rimane uno dei problemi più sentiti da tutti i nostri cittadini. Insomma, un vero disastro, sotto tutti i punti di vista. Recenti vicende, come la crisi finanziaria di Taranto o il ripiano dei debiti sanitari delle varie Regioni in discussione oggi, chiaramente anticostituzionale (è stato deciso con decreto in questi giorni), ripropongono con forza un'annosa questione. Deve o non deve il Governo centrale intervenire per salvare un governo locale in crisi finanziaria irreversibile? La nostra stessa Costituzione sembra escluderlo, tant'è che all'articolo 119 recita: «È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti» (dagli enti territoriali). Ma la risposta onesta è che in molti casi lo Stato non può farne a meno, per la presenza di altri vincoli costituzionali, non meno pregnanti, e di proprie specifiche responsabilità nella vicenda. Ma azioni di salvataggio possono generare aspettative pericolose di *bailing out* generalizzato per tutti gli enti locali, con il rischio di scatenare un'irresponsabilità finanziaria diffusa. È perciò necessario che questi interventi, quando si fanno, siano accompagnati anche da forti sanzioni per gli enti locali coinvolti, che incidano sugli amministratori, sui cittadini stessi, "colpevoli" di aver eletto dei governanti incompetenti. Per i politici locali, la sanzione ultima non può che essere la soppressione della propria sovranità, almeno per un tempo determinato; per non parlare della parte politica che sostiene questo sistema sanitario: sì alla droga, bocciato sonoramente da una sentenza del TAR. Si chiudono i laboratori privati; si lascia la gente in coda ai CUP per una prenotazione che avviene tra i sessanta e i Si va in giro per convegni, ma in giro per gli ospedali finora quasi nulla. Questo è il Governo dei colpi di spugna, che proprio la Turco ha avallato, come, ripeto, gli esempi delle Regioni che stiamo trattando. Non è questa la sanità dei cittadini. Questo è il disservizio sanitario a carico dei cittadini che, ricordiamolo, sono i primi contribuenti. Oggi, cari colleghi, dobbiamo votare in Aula un provvedimento anticostituzionale. Prima di esprimere il nostro voto, facciamo una seria riflessione. *(Applausi del

sanità a livello nazionale, che hanno visto anche i Governi precedenti impegnati a dare una mano seria e sostanziale alle Regioni con situazioni pesanti dal punto di vista finanziario.

Per la posizione che assumiamo rispetto a queste vicende regionali dobbiamo far presente all'Aula e ai colleghi senatori che in alcune situazioni regionali abbiamo a che fare con una sanità che fare con una sanità pubblica che sostiene strutture importanti dal punto vista del Servizio sanitario nazionale, con finanziamenti che già in passato erano stati consistenti e che hanno continuato ad essere giustamente erogati, perché credere in un Servizio sanitario nazionale significa poi sostenerlo.

e negli anni passati hanno avuto anche un grande slancio in termini di ripresa e di sviluppo: basterebbe soltanto esaminare i bilanci regionali e verificare

è accreditato e convenzionato esso svolge una funzione sostanzialmente pubblica a favore dei cittadini. Quindi, anche in questo senso occorre tener presente che tali bilanci risentono di un di un intervento finanziario a favore di queste strutture, che in passato hanno provocato altri interventi da parte di Governi precedenti che oggi si muovono in questa direzione. *(Brusìo).* PRESIDENTE. Colleghi, c'è un disturbo continuo. Senatore Procacci, sta parlando il senatore Cursi: lo guardi quando parla. Mi scusi, senatore importanti da sostenere a livello nazionale, così come importanti sono le strutture delle altre Regioni, che non sono comprese nel piano di intervento di questo decreto-legge che oggi stiamo esaminando. Ciò posto, mi consenta l'Aula di sostenere anche Leggendo il decreto-legge verifichiamo che a fronte dei disavanzi che presentano le Regioni è richiesto un piano di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale diretto alla riduzione strutturale della spesa e al perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario corrente.

basterebbe immaginare che è partito lo scorso anno e che faceva parte degli accordi già fissati dal precedente Governo Berlusconi e dall'allora ministro Storace, quando i piani di rientro dovevano essere effettuati essere effettuati seguendo certe logiche e certe procedure. Bene, la Regione Lazio ci ha messo ben otto mesi circa, quindi vuol dire che qualcosa non funzionava, vuol dire che spesso questi piani di rientro erano soltanto impegni di carattere generico non suffragati e non sostenuti. Così come

non è sostenuto dal punto di vista della certezza su dati di fatto incontrovertibili, cioè è venuta fuori l'inattendibilità di questi dati, è venuto fuori, dal

delle Commissioni riunite, quegli elementi di certezza che ci diano la possibilità di stabilire con certezza lo sbilancio complessivo della Regione Lazio. Vediamo però che la stessa Regione

presenta una situazione di sbilanciamento che sicuramente non va nell'ottica del rientro e, come dice la legge, della riduzione strutturale della spesa e del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, se nel 2006 il Lazio presenta 1,4 miliardi di sbilanciamento. Ciò vuol dire che il piano di risanamento non viene perseguito, vuol dire che la cultura che tende a ridimensionare la spesa non c'è, vuol dire che alcuni fatti che stanno avvenendo anche a livello della Regione depongono in maniera contraria. Cito un paio di

dagli IFO oncologici, San Gallicano e Regina Elena. Com'è possibile spiegare all'opinione pubblica, sul piano del contenimento della spesa, che si chiude un centro trapianti si chiude un centro trapianti al Regina Elena, un centro trapianti e un ospedale che sono a livelli eccezionali dal punto di vista della qualità dei servizi, e poi si fa il primo trapianto nei giorni scorsi nella sala di cardiochirurgia del San Camillo? Poi leggiamo

Ho avuto occasione già di dirlo nelle Commissioni riunite e lo ripeto in questa sede: noi vorremmo che, accanto a questa operazione (nei confronti della quale abbiamo già preannunciato in Commissione, e riconfermiamo in questa sede, il nostro voto di astensione),

se è vero che le vicende legate al piano rifiuti della Campania stanno creando grossissimi problemi da un punto di vista sanitario e, in quel contesto, la sanità paga, quindi è in quel contesto che vengono stanziati i soldi all'interno di un piano sanitario regionale.

Che dire poi della spesa per i medici assunti oggi con contratto a tempo determinato quando, rispetto agli specializzandi, sempre nei piani di rientro - perché anche questi costano

di sottoscrivere un'interrogazione che potesse affrontare il tema degli specializzandi in maniera seria; e il Gruppo di Alleanza Nazionale, in maniera seria, sottoscrisse quella interrogazione. Ebbene, ad oggi ancora non si è fatto nulla; gli specializzandi sono ancora senza un trattamento serio

che il dibattito di oggi serva anche ad affrontare questi temi, ma soprattutto ad affrontare il tema serio di come spendere i soldi pubblici, che mettiamo a disposizione anche con questo decreto-legge. Se così non facessimo,

non solo attraverso l'accompagnatore di turno, di affrontare alcune tematiche e di intervenire in maniera seria anche attraverso sanzioni di carattere amministrativo nei confronti delle Regioni

Signor Presidente, la conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, evidenzia molteplici contraddizioni politiche e soprattutto palesa incomprensibili atteggiamenti che nel rapporto Stato-Regioni finisce con il discriminarne alcune a danno di altre, promuovendo quelle Regioni meno virtuose che hanno finito con l'accumulare notevoli disavanzi nel periodo 2002-2005. Nel decreto-legge si evidenzia in più riprese che trattasi di un intervento assolutamente eccezionale e straordinario che offre una via d'uscita per il risanamento e il rilancio dei servizi sanitari che nelle Regioni interessate si troverebbero altresì in condizioni drammatiche, con pesanti conseguenze per i cittadini. Ci si accinge con questo provvedimento - è detto - ad erogare finanziamenti a Regioni che hanno accumulato negli anni debiti consistenti, costringendole (si fa per dire) ad un accordo obbligatorio, di certo non chiaro e tanto meno concretizzato, sul piano del rientro e ad adottare misure per la riorganizzazione del sistema sanitario. È davvero difficile - mi consenta, signor Ministro - comprendere la logica ispiratrice dell'azione di Governo in tutto questo, che, anziché riconoscere l'imprescindibile equità di giudizio, per cui tutte le Regioni sono uguali dinanzi alla legge, ricorre a criteri selettivi per regolare l'accesso ai 3 miliardi di euro delle Regioni in disavanzo. Appare di gran lunga, infatti, un criterio ambiguo, che finisce con l'attribuire una scarsa ricompensa a coloro che hanno mantenuto una situazione di sostanziale equilibrio e premia invece, in maniera sproporzionata, con incentivi, chi ha male amministrato e creato debiti astronomici a volte ben mascherati. Esiste una chiara violazione del principio di uguaglianza stabilito, peraltro, dalla Costituzione. Lo stesso titolo del decreto evidenzia in forma palese tutto questo: parla di «ripiano selettivo» dei disavanzi pregressi e ciò evidenzia palesi discriminazioni. Si tratta di una profonda lesione del principio di uguaglianza e della ragionevolezza, che vorrebbe non un criterio selettivo, ma un criterio equo nella ripartizione dei fondi nazionali. Allora, perché ricorrere ad un decreto d'urgenza per ripianare disavanzi che, tra l'altro, non sono recenti ma datati 2002-2005? Perché - ci domandiamo - lo Stato deve intervenire con un provvedimento volto a sanare l'inefficienza cronica di alcune Regioni e che rischia, nel complesso, di compromettere e disincentivare successivamente l'azione di altre Regioni cosiddette virtuose dal perseguimento dell'obiettivo del buon andamento dell'amministrazione? Non è equo tutto questo; anzi, è falsamente solidale ed ingiusto consentire che l'accesso ai 3 miliardi straordinari di euro disponibili sia riservato soltanto ad alcune Regioni, ripeto, quelle meno virtuose, mentre le altre, non avendo accumulato disavanzi o avendo in maniera tempestiva provveduto con risorse proprie alla predisposizione di piani di rientro, si vedono danneggiate da un simile provvedimento. Sia chiaro, noi non avremmo di certo auspicato che il risanamento dei conti pubblici si fosse concretizzato con tagli indiscriminati alla spesa sanitaria, alle prestazioni o ai posti letto ospedalieri, ma avremmo apprezzato di più e plaudito persino all'azione di un Governo che avesse spinto con più coraggio le Regioni, più coraggio nel determinare e nel pretendere la qualità, l'appropriatezza della spesa e l'allocazione delle risorse. Avremmo voluto che fossero resi ben più chiari e trasparenti i controlli della spesa relativi agli appalti, alle convenzioni, alle esternalizzazioni. Avremmo voluto più chiarezza da parte delle Regioni nell'assunzione di impegni certi, visto tra l'altro che l'80 per cento dei bilanci regionali è destinato alla sanità. Ma in questo decreto, purtroppo, di tutto ciò non c'è nemmeno una traccia, nemmeno una garanzia e tanto meno compare la cancellazione di quella preoccupazione, convitata di pietra a questo dibattito, che, per sanare debiti pregressi, se ne creino di nuovi. Non vorremmo, infatti, assistere ad un consolidamento cronico del debito, incrementato a dismisura da politiche sanitarie confuse, contraddittorie e per questo dannose. L'azione del Governo avrebbe avuto un senso - parliamoci chiaro - se fosse stata commisurata in parallelo o successivamente all'adozione da parte delle Regioni interessate di una serie di accorgimenti e di sistemi volti a garantire un serio impegno e a far sì che le risorse non fossero sprecate e tantomeno i pazienti trasformati in una sorta di bancomat da spennare per ripianare gli sprechi. La riforma del Titolo V della Costituzione ha sostanzialmente modificato i rapporti Stato-Regioni nella gestione del servizio sanitario suddividendo in forma netta oneri e responsabilità; responsabilità che, in fatto di copertura degli eventuali disavanzi di gestione, sono attribuite in forma chiara alle Regioni. Non è quindi pleonastico affermare che si tratta di un'ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali. Siamo in presenza di una sovrapposizione di politiche governate centralmente rispetto a quelle che legittimamente dovrebbero essere decise dalle Regioni. Ora con questo provvedimento si stabilisce un nuovo criterio, quello cioè della sovrapposizione di ingiustificabili operazioni statali di ripiano destinate, per certi versi, a scoraggiare la voglia di risanamento dei conti regionali e, per altri, addirittura ad indebolire le aspettative delle Regioni virtuose circa la serietà del patto stipulato o stipulabile con lo Stato. Come fare in questa ottica a non considerare come fondato il sospetto di una disparità di trattamento tra Regioni che in questo contesto rischiano di essere divise tra Regioni amiche e Regioni più amiche? È davvero contraddittorio il comportamento di uno Stato che, nel mentre mantiene l'iniquo *ticket* di 10 euro a ricetta sulle prestazioni diagnostiche e specialistiche, non riuscendo a trovare 811 milioni di euro che sarebbero necessari per la sua soppressione, tempestivamente però riesce a tirare fuori dal cilindro addirittura 3 miliardi di euro per ripianare i disavanzi pregressi delle Regioni meno virtuose. Parimenti e su questa linea non condividiamo affatto la scelta di non avere previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la percentuale minima delle ulteriori risorse che devono essere destinate alla sanità in via aggiuntiva rispetto all'innalzamento delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP ai massimi livelli per le Regioni che accedono al riparto dei 3 miliardi di euro. Potrebbe infatti accadere che accedano al finanziamento straordinario statale anche Regioni che, pur in presenza di ingenti disavanzi, ricorrono in maniera minima all'innalzamento della leva fiscale. Se la spesa sanitaria di alcune Regioni è rimasta fuori controllo le responsabilità vanno individuate, non occultate, oltre che nelle modalità in cui si articola la spesa regionale, anche nell'assoluta mancanza di sistemi di controllo e verifica sia nell'erogazione che nel costo della prestazione sanitaria, nell'errata previsione della spesa, nelle lacune di una programmazione nazionale e regionale fondata, oltre che su dati epidemiologici certi, sulle effettive necessità del cittadino sul territorio. In molte Regioni i sistemi di controllo e verifica non hanno mai, o quasi mai, funzionato in maniera corretta; non si è operata una vera razionalizzazione delle risorse e della rete sanitaria, volta ad eliminare gli sprechi e a liberare risorse per consentire il miglioramento della qualità assistenziale del servizio sanitario. Uno sguardo complessivo sul modello di sanità italiana non può non rilevare l'esistenza di un servizio sanitario che spesso, in fatto di qualità, si configura a cosiddetta macchia di leopardo, con ospedali - ad esempio, quelli presenti in alcune Regioni del Centro-Sud - che somigliano, a detta persino di coloro che vi operano, a dei veri e propri gironi danteschi dove, nonostante la dedizione di alcuni, gli operatori sanitari sono costretti a sopravvivere tra mille difficoltà, risorse insufficienti o malamente assegnate. Si giustifica davvero poco, che sia l'intera collettività a ricoprire, ancora una volta, il costo dell'inefficienza dell'incapacità gestionale di alcune amministrazioni regionali che, per demagogia, non introducono il *ticket* sui farmaci, per esempio, pur essendo consce che la spesa farmaceutica rappresenta la principale fonte di sfondamento dei bilanci sanitari. Ciò che oggi più di tutto chiede il Paese è un credibile governo dei servizi sanitari, un governo capace di soddisfare efficacemente la domanda al bisogno di assistenza. Ma per fare questo non ci può accontentare di un tirare a campare, perché in sanità questo rischia di trasformarsi in un tirare le cuoia. Occorre qualificare allora la spesa, tagliare gli sprechi, sanare l'uso distorto delle risorse ed eliminare, soprattutto, le sacche di inefficienza. Sicuramente, quanto fatto dal Governo con questo decreto non è educativo e tantomeno equo. Insinua semmai il sospetto e la diffidenza che, pur in assenza di un ravvedimento, si sia voluto offrire, a spese di tutti i di tutti i cittadini, il vitello grasso in onore del figlio, *pardon,* di alcune Regioni predilette, escludendo però dal tavolo dei commensali coloro che invece hanno dimostrato serietà, affidabilità e lealtà. È imperdonabile un simile colpo di spugna sulle responsabilità acclarate, che finisce con una paradossale finzione: quella di ammettere, nella notte senza stelle, che tutte le mucche sono nere e tutte le Regioni sono uguali, senza discrimini tra quelle virtuose e quelle che non lo sono. Sono tutti questi interrogativi, in sintesi, che ci lasciano senza convincenti riposte, a motivare la nostra contrarietà alla conversione in legge di questo decreto riguardante il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario.

ricorrere a ripianare debiti delle aziende sanitarie locali. Ricordo che qualche anno fa - era allora presidente del Consiglio l'onorevole D'Alema ci fu un attento dibattito in Parlamento sul tema del ripiano dei debiti delle unità sanitarie locali, quindi delle Regioni. In quel momento discutemmo anche del ripiano dei debiti del Policlinico Umberto I. Desidero, quindi, richiamare l'attenzione del Ministro della salute,

in questi giorni è stata emanata una circolare del direttore sanitario di quell'azienda, il dottor Dal Maso, che mette a disposizione del DEA di secondo livello, quindi del pronto soccorso di quella struttura ospedaliera, 1.300 giovani medici specializzandi che operano nel Policlinico Umberto I, nella più importante facoltà di medicina d'Italia. Ieri sera l'ho voluto ricordare

famosa, l'ospedale Sant'Andrea; fu necessaria la Giunta di centro-destra alla Regione Lazio per aprire, dopo 27 anni, l'ospedale Sant'Andrea. Ma non è tutto: ci vollero i fondi della regione Lazio per aprire e mettere in funzione uno dei più bei policlinici universitari d'Italia: il Policlinico di Tor Vergata. Invece, nel progetto di ripiano della Regione Lazio, vi è stato l'accordo stipulato dal presidente Marrazzo con il ministro Padoa-Schioppa. E guarda caso,

la cancellazione di strutture ospedaliere del centro della città di Roma. Si parla della chiusura del Nuovo Regina Margherita, che è ormai una cosa conclusa perché si stanno già spostando i reparti, ed anche della chiusura di una struttura ospedaliera vicina

Mentre ciò avviene, il direttore generale dell'azienda San Camillo-Forlanini acquista una nuova TAC per l'ospedale Forlanini, che viene contemporaneamente messo in disuso, per oltre due milioni e mezzo di euro,

dopo alcuni mesi, a nominare il direttore generale di un'azienda importante come l'azienda sanitaria di Latina. Questo avviene anche perché ultimamente i direttori generali che furono cacciati quanto nominati dalla Giunta Storace, e che non avevano raggiunto il periodo del contratto, hanno vinto prima il ricorso al TAR e poi addirittura al Consiglio di Stato. Quindi ci troveremo nella situazione - forse il Ministro non lo sa che in cinque ASL la Regione Lazio dovrà pagare lo stipendio di almeno due direttori generali, perché i direttori generali che hanno vinto il ricorso sono nella possibilità di riprendere il loro ruolo o di contrattare con la Regione una buona uscita che verrà a pesare ulteriormente

motivo nell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I si devono utilizzare i giovani medici? Perché ai giovani medici non saranno pagati - la legge lo prevede - i turni che effettueranno al pronto soccorso e al DEA di II livello. si verifica una situazione paradossale: i giovani medici che entrano in servizio e saranno i facente funzione delle attività del Policlinico non saranno pagati, mentre il direttore generale Montaguti si è aumentato lo stipendio di un altro 30 cento. Se vogliamo arrivare ad una situazione complessiva che ci permetta di guardare realmente alla spesa di questa Regione, penso alle iniziative che hanno portato avanti

alla Regione il pagamento dei loro crediti per due anni. Cosa avviene? Quello che è stato denunciato sulla stampa romana e laziale, cioè si rischia di mandare a casa decine e decine di piccole aziende che sono fornitrici ufficiali delle aziende sanitarie della nostra Regione. Come si fa il risanamento?

dell'agenzia di sanità pubblica parla di una cifra di diminuzione di posti letto, mentre l'assessore alla sanità ne dice un'altra; poi il presidente della Regione Marrazzo dice che va a inaugurare i cantieri al Policlinico, quando - interpellato da me - il Rettore Magnifico dell'Università di Roma sostiene che non c'è alcun cantiere all'interno dal Policlinico Umberto I. Allora si sta giocando sulla pelle dei cittadini e quei cittadini del Lazio Alleanza Nazionale li sosterrà nella battaglia contro la chiusura degli ospedali di questa città. *(Applausi

sbagliato e ciò almeno per tre ordini di motivi: il primo riguarda le regole, il secondo riguarda la Costituzione e il terzo le modalità dell'accordo tra Stato e Regioni in materia. Per quanto concerne

Si tratta, ovviamente, di un'opera molto difficoltosa che può essere esperita con il passare del tempo e con il miglioramento delle tecniche di controllo e di spesa, ma che, in ogni caso, non può essere abbandonata.

si sono comportate in modo per loro svantaggioso, che, alla fine, interviene sempre lo Stato a finanziare *a posteriori* anche gli sfondamenti delle Regioni meno virtuose.

ha posto in essere azioni serie di contenimento della spesa sanitaria, mentre adesso, proprio ultimamente - forse è cambiata anche la maggioranza politica invertito completamente la sua rotta, iniziando a spendere in modo molto pesante e si presume che prossimamente vada al di là degli obiettivi. Ciò significa che fino a quando esiste una guida seria della finanza pubblica in questo settore, la spesa viene contenuta; quando invece questa guida viene meno, la spesa inizia travalicare. Ciò significa tra l'altro che, se così si procederà nel futuro, la spesa sanitaria crescerà in modo esponenziale e sarà difficilissimo riporla sotto controllo, anche perché l'aspetto emulativo verrà meno. La seconda questione, ed è una questione molto rilevante che credo riguardi anche la Presidenza del Senato, è che il decreto-legge in questione non si limita a fissare dei meccanismi relativamente alla copertura dei disavanzi, segnatamente nel primo comma, e quindi a rendere automatici dei meccanismi di inasprimento delle sovraimposte delle aliquote fiscali, ma opera una sanatoria *a posteriori* del debito, sostanzialmente finanziando con 3 miliardi di euro il debito pregresso delle Regioni. Ciò, e mi meraviglio francamente che il Presidente della Repubblica abbia firmato questo decreto, decreto, contravviene espressamente con l'ultimo comma dell'articolo 119 della Costituzione, che recita: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese d'investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato su prestiti dagli stessi contratti». Questo significa che non è possibile indebitarsi

di 3 miliardi di euro autorizzata da questo decreto è chiaramente contraria all'articolo 119 della Costituzione. Mi domando come ciò sia stato possibile, tenendo conto che il decreto è passato attraverso il vaglio della Presidenza della Repubblica.

e di altri soggetti, facendo caducare una norma posta dal legislatore costituzionale nel 2001 a salvaguardia della finanza pubblica, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di Maastricht. Tra l'altro, vale la pena far presente che se tra i vari obiettivi di finanza pubblica definiti a livello europeo, insieme a quelli di carattere quantitativo relativi all'attuazione dell'ultima manovra finanziaria, l'attuale Governo aveva posto anche quello delle cosiddette riforme strutturali, nel momento in cui, in un settore così importante della finanza pubblica, come la spesa sanitaria, esso rinuncia a qualunque tipo di controllo della spesa e va verso un lassismo inconsiderato, da chiedersi come questo possa conciliarsi con gli obiettivi assunti dal Governo e dal Ministero dell'economia - il sottosegretario Sartor dissente, ma mi permetto di chiedergli

La terza questione concerne l'accordo con le Regioni. In questa materia si è sempre cercato un accordo con le Regioni per definire le modalità di suddivisione della spesa sanitaria

-, ma faccio presente che due Regioni hanno già impugnato presso la Corte costituzionale il decreto medesimo. Mi domando, in ogni caso, ha senso recepire acriticamente un accordo con le Regioni, anche quando questo anche quando questo viene fatto in violazione di una norma costituzionale? Credo che il Parlamento abbia in ogni caso il diritto e il dovere di valutare,

tutti i soldi soltanto ad alcune Regioni e far sì che sostanzialmente non vengano smussate le situazioni di iniquità

decreto-legge una sorta di fonte normativa atipica e quindi da approvare nella sua totalità perché atto sottoposto ad un preventivo accordo accordo e quindi non modificabile, ma a entrare nel merito del contenuto dell'accordo per modificarlo laddove ciò sia indispensabile. Questa è la sintesi delle osservazioni relative al provvedimento in esame, tenendo conto che esso è criticabile, a mio sommesso avviso, e non corrisponde ai criteri di costituzionalità. Pertanto, andrebbe ampiamente corretto

Saluto, a nome dell'Aula, i giovani della scuola media «Zingarelli» di Foggia che seguono i nostri lavori dalle tribune.

La legge finanziaria per il 2007 (all'articolo 1, comma 796, lettera *e)* consente alle Regioni che presentano un *extra-deficit* nel settore sanitario, di sanare i disavanzi pregressi, registrati fino a tutto il 2005, mediante una copertura pluriennale. A tal fine viene prestato il concorso dello Stato (e quindi della comunità nazionale dei cittadini)

della leva fiscale (ancora una volta quindi a carico della comunità regionale in questo caso) ovvero la destinazione alla copertura delle perdite sanitarie di entrate tributarie che attualmente finanziavano altre funzioni di spesa, (e quindi sottraendo altre risorse alla comunità regionale dei cittadini). Ho analizzato nel merito la norma che ha consentito il decreto-legge che stiamo discutendo per arrivare a fare una valutazione: sostanzialmente questo progetto di ripiano mette a carico dei cittadini l'intero costo della manovra, che per quanto riguarda l'intervento dello Stato, è pari a circa tre miliardi di euro. E sulle cause e le responsabilità di questo disastro, quali risposte abbiamo tutti insieme individuato? Il relatore in Commissione, il collega Tecce di Rifondazione Comunista, ragionando parlava di due cause: da un parte di cattiva gestione della politica sanitaria e, tra le altre, diceva anche che sicuramente vi è un ragionamento che coinvolge il punto delle politiche del malaffare. Queste erano le due cause che individuava. uscendo dalla genericità semplicistica, nelle due Regioni più significativamente toccate dal provvedimento - mi riferisco al Lazio e alla Campania - quali concrete patologie sono state individuate? Noi non potremo mai curare una malattia se non ne indichiamo con precisione la natura e le cause.

per evitare di essere considerato fazioso e portatore di conflitti per reticenza interessata, preferisco essere ancora più chiaro, occupandomi della Regione nella quale vivo (la Campania) e tralasciando il Lazio, del quale (a parte i recenti scandali emersi sui *media*) poco conosco del merito tecnico-gestionale. In Regione Campania, onorevoli colleghi senatori, abbiamo un assessore alla sanità "esterno" (il dottor Angelo Montemarano) il quale pur essendo continuamente impegnato per le varie campagne elettorali, anche congressuali - dal 2005, quindi da circa due anni si sta occupando anche del ripiano del *deficit* sanitario di quella Regione. Devono sapere i colleghi che buona parte di tale *deficit* per la Campania (forse in una misura che potremmo quantificare ben oltre il 30 per cento) proviene dalla più grossa Azienda sanitaria locale, la Napoli 1,

che fino a due anni fa era governata dallo stesso Montemarano che, giusto per dirla tutta, è stato direttore sanitario, sempre della ASL Napoli 1, dal 1996 al 1998, per diventarne poi il direttore generale dal 1998 fino al 2005, quando è diventato

possa poi curarla o che, usando una metafora diversa, chi ha commesso il reato poi cerchi di individuare i colpevoli e le responsabilità? Mi sorprende che gli amici di Rifondazione Comunista, pur conoscendo i fatti, pur avendo fatto in Regione mille battaglie, tutte lodevoli e apprezzabili, su questo punto siano leggermente distratti, perché non approfondire questa tematica determina purtroppo il perpetrarsi di errori dannosi per il nostro Sud. In Campania, Presidente, il *deficit*, oltre che dalla spesa farmaceutica, che determina un disavanzo che potremmo quantificare intorno al 18-19 per cento, nasce anche dalla circostanza che non esiste ancora alcuna forma controllata di accreditamento delle strutture private, il che determina una spesa assolutamente non prevedibile, non programmabile, non controllabile e quindi senza limiti.

perché con l'accreditamento provvisorio si evitano i controlli che dovrebbero determinare la chiusura delle strutture non a norma e pericolose e perché nella provvisorietà senza regole il potere discrezionale è più ampio e consente maggiore arbitrio e più abusi, e quindi un ritorno elettorale ancora maggiore. Questa è la situazione più grave che incide direttamente sul *deficit*

finanziario internazionale. Penso di avere reso il mio pensiero; riduco il mio intervento in omaggio alle pressioni del Presidente. Non voglio dilungarmi, però questa cura sperimentale di ripiano è costosissima e pericolosa. Mi rivolgo al Ministro:

Sto concludendo, grazie. È molto difficile, capisco che si tratta di argomenti un po' ostici per tutti, Presidente, ne prendo atto. PRESIDENTE. No, questo non glielo consento:

Allo stato, devo purtroppo affermare che è molto difficile condividere responsabilità che, senza risolvere i problemi e senza garantire un servizio sanitario efficiente, di fatto continueranno a favorire il malaffare. Io non voglio essere corresponsabile di ciò. Presidente, in realtà il collega Manzione, parlando della sanità in Campania,

soffermarmi su tre questioni, avendo ascoltato il dibattito. Da una lettura attenta del provvedimento dalla contestualizzazione dello stesso nell'ambito della politica sanitaria che il Governo sta portando avanti

che nella fase applicativa dei piani di rientro sia coinvolto il Parlamento. Noi sentiamo l'importanza di condividere questa difficile e impegnativa azione di efficienza del sistema sanitario non soltanto con le Regioni ma con l'insieme del Parlamento, perché la sfida è proprio questa: mettere sotto controllo la spesa sanitaria del nostro Paese e farlo in quelle Regioni che, nel corso di tanti anni, hanno accumulato debiti pesanti, debiti che, nel patto per la salute, nella legge finanziaria di cui questo è decreto applicativo, si stabilisce che debbano essere estinti entro il 2010. Quindi vorrei rassicurare il senatore Manzione e dirgli che l'impegno di questo decreto attiene al rendere effettivo quanto stabilito nella finanziaria,

l'efficienza della spesa sanitaria, nella consapevolezza che l'efficienza è l'altra faccia dell'equità, che l'efficienza è sostanziale per promuovere il dritto alla salute. Vi è anche un altro elemento che è alla base di questo provvedimento: mi riferisco alla promozione dell'unitarietà del sistema, in quanto noi siamo per un federalismo solidale. Siamo per un federalismo solidale perché la tutela del diritto alla salute, sia attraverso il contenimento delle liste d'attesa, sia per promuovere le politiche di prevenzione, sia per estendere i centri di eccellenza, ha bisogno di un sistema sanitario unitario; un federalismo solidale, ed è questo l'intento del provvedimento, che abbia come obiettivo di far sì che tutte le Regioni, dal Lazio alla Sicilia, entro il 2010 azzerino i loro debiti. Ripeto, questo è l'intento del provvedimento:

della strumentazione normativa che si pone come sviluppo dei patti di stabilità e di contenimento della spesa avviati dai Governi precedenti, tant'è che noi li richiamiamo. Vi è però una novità

la strumentazione che è stata messa in atto nella finanziaria consentirà al Governo di controllare l'applicazione dei piani stessi. Noi controlleremo tale applicazione. La norma contenuta nella finanziaria di fatto prevede da parte delle Regioni che hanno pesanti debiti una cessione di sovranità.

controllo dell'accreditamento tra pubblico e privato, promozione della medicina territoriale. Se leggerete i piani di rientro - io sarò felicissima di poterli consegnare al Parlamento - noterete che sono contenuti indirizzi molto severi

quindi una cessione di sovranità e io propongo in quest'Aula, come ho fatto in Commissione, che il controllo sull'attivazione dei piani di rientro sia esercitato anche dal Parlamento. La posta in gioco è grandissima ed è la tenuta del sistema sanitario pubblico, universalistico e solidale, perché sappiamo bene che il diritto alla salute significa avere le garanzie che le risorse stanziate siano

condividiamo il principio, però, come sapete, non è tecnicamente praticabile perché implica una separazione, all'interno del bilancio regionale, che è unico, delle voci correlate e delle spese per la salute.

una raccomandazione per il futuro perché noi siamo per il federalismo fiscale, ci stiamo lavorando. *(Commenti dal Gruppo LNP)*. Siamo per il federalismo solidale che significa prevenire le situazioni debitorie.

con le Regioni, che aumenta di 6,5 miliardi, dal 2006 al 2007, le risorse per i livelli essenziali di assistenza; prevede risorse certe, sempre per i livelli essenziali di assistenza, per i prossimi tre anni,

In Campania - hanno ragione alcuni colleghi del centro-sinistra - si verifica un malgoverno della sanità che è quasi familistico, perché siamo arrivati al punto che l'assessore regionale alla sanità, il dottor Montemarano, è stato anche promotore della candidatura

ingiusto che i cittadini campani debbano fronteggiare 3 miliardi di euro di *deficit* della sanità, soldi che sono stati anticipati per il ripianamento delle perdite dalla Morgan Stanley, una banca che vede al suo interno tra i funzionari di primo piano il figlio del Presidente della Regione Campania. Montemarano gestisce la sanità in funzione di aggregati parentali e la stessa cosa avviene per quanto riguarda la gestione del debito. Tutto ciò è il segnale di come in quella Regione si sia

Credo che in qualche modo lei debba prendere delle misure nei confronti di questo senatore maleducato, come minimo, della cui intelligenza

il Gruppo di Alleanza Nazionale ha osservato l'*iter* di questo decreto-legge con l'attenzione che merita, senza stupirsi molto rispetto ai contenuti. è un passo avanti molto importante rispetto alla propaganda che si fa fuori dalle Aule del Parlamento quando si dice che si ha un nome e un cognome nella responsabilità del debito della Regione che mi è capitato di governare per volontà popolare. Questo lo considero un passo avanti. Qual è il problema che ci impedisce di sostenere un decreto del genere? Prego il collega Cursi di farmi parlare con il Ministro, perché vorrei avere attenzione rispetto agli argomenti. Vede, signor Ministro, se si fa propaganda attorno a un decreto-legge poi è difficile trovare un punto d'intesa. Allora è necessario che si abbia l'onestà di dire al Parlamento quali sono i problemi strutturali delle Regioni, e di alcune Regioni, perché ad esempio la sanità della Regione Lazio (lo voglio fare con lo stesso spirito di onestà intellettuale del collega Manzione nei confronti della sua Regione) ha un problema che precede e segue la mia stessa amministrazione regionale. Lo voglio dire anche ai colleghi degli altri Gruppi dell'opposizione, di cui rispetto la libertà di voto, ci mancherebbe altro. Ci sono stati molti assessori alla sanità in questa Regione: penso a quelli che precedettero la mia amministrazione, allora erano Partito Comunista, poi diventati Democratici di Sinistra; penso a quelli che hanno accompagnato la mia amministrazione, il Gruppo Forza Italia; penso a quelli che ci sono adesso.

e ciò significa anche la possibilità di impiegare la migliore gioventù del Paese. È una Regione, quando parliamo di sanità privata, che ha una proliferazione di sanità religiosa, la cosiddetta classificata; è quella, colleghi, che attrae malati da tutte le Regioni d'Italia. Signor Ministro (mi dispiace che non riesca ad ascoltare, vorrei che avesse un po' di attenzione verso chi l'ha preceduta nel suo incarico, perché magari su alcune questioni ci si può intendere), lei ha ragione quando dice che la regola che sta nel decreto viene esattamente dalla regola che introducemmo, su mia proposta, nella finanziaria del Governo Berlusconi, scritta con i colleghi Vegas e Tremonti,

Però lei, signor Ministro, ci deve aiutare ad avere chiarezza su questo *bluff* dei conti, perché sulle carte che lei ha portato qui (ed è questo l'errore, collega Polledri, nell'ordine del giorno), in nessuna parte si parla di 10 miliardi; di più: si parla di 2 miliardi di crediti, e non di debiti, che la Regione deve avere dallo Stato, si dimezza sostanzialmente il disavanzo dividendolo in parte tra l'amministrazione che è toccato presiedere a me e quella attuale, perché parliamo di quasi 3 miliardi di euro per il 2005-2006.

di diverso rispetto alla nostra amministrazione? Si è rinunciato al *ticket* sulla farmaceutica, si è rinunciato alle alienazioni degli ospedali pubblici, si sono transati fondi ingenti con i privati che hanno contribuito ad aumentare il disavanzo della Regione Lazio. Questa è la realtà di oggi.

la sua copertina, hai voglia a parlare dell'eredità! Gli strofinacci al presidente Marrazzo glieli abbiamo lasciati, ma il Policlinico versa nell'immondizia e nel degrado. Sono questioni che lei, signora Ministro, ha il dovere di sollevare con forza nei confronti della nuova amministrazione regionale, altrimenti non serve venire in Parlamento. Rivolgendomi ai colleghi degli altri Gruppi della minoranza, ricordo che questi decreti li abbiamo approvati anno dopo anno.

Per troppo tempo si è cianciato di sanità privata. Lo voglio dire a chi fa lo spiritoso su certi episodi che nel Lazio sono stati fortunatamente scoperti, mentre in altre Regioni non sono stati neppure cercati. Questa è la verità, perché la sanità privata sta dappertutto. io posso vantare un orgoglio. Quando oggi si parla di sanità, in tutta Italia posso trovare tre strutture ospedaliere in più: l'Istituto tumori, il Policlinico di Tor Vergata e il Policlinico Sant'Andrea. Questa, colleghi, è sanità pubblica, non privata.

tra Stato e Regioni che giustifica la necessità di un'attenta valutazione, visto che spesso la Corte costituzionale ha dato ragione alle Regioni e torto allo Stato. Quindi, chiediamo al Ministro di accogliere una

testo riformulato, e del senatore Calderoli sia esattamente all'interpretazione letterale dell'articolo 119 che, come è noto, prevede le risorse aggiuntive per le aree sottoutilizzate.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.47,

1.539, 1.540, 1.544 e 1.0.4. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti

Esprime quindi parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.0.200 sul quale il parere è rinviato». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.0.200 ed i relativi subemendamenti 1.0.200/1 e 1.0.200/2, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sull'emendamento 1.0.200 e sul subemendamento 1.0.200/1 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 1.0.200/2». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.505 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea e relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario».

che in quest'Aula rappresentano collegi, territori e Regioni che negli anni hanno intrapreso una politica di rigore nella gestione del sistema sanitario, anche attraverso l'inserimento di aliquote aggiuntive (IRPEF e IRAP) e in alcuni casi con considerazioni significative, come il concetto di compartecipazione

che negli anni hanno proceduto, nei confronti dei loro cittadini, ad inserire elementi di compartecipazione per finanziare i disavanzi sanitari, oggi si vedono superate da un provvedimento che le esclude totalmente dalla suddivisione di questo stanziamento. Beninteso, non sono contrario allo stanziamento, perché conosco bene la situazione debitoria delle Regioni, ma credo che il sistema adottato - e con questo emendamento proponiamo un meccanismo diverso di destinazione delle risorse delle risorse - sia iniquo per i motivi di carattere costituzionale che dicevo poc'anzi, ma soprattutto per questioni di modello. Infatti, cosa evinceranno le Regioni nel momento in cui questo provvedimento verrà approvato? che non devono più procedere attraverso l'impegno personale sul proprio territorio, ma semplicemente aspettare, come sempre è stato fatto, che il Governo ad un certo punto stanzi delle risorse per ripianare i loro debiti.

Ebbene, questo provvedimento fa cadere qualsiasi elemento di responsabilità da parte delle Regioni, demandando, ancora una volta, il concetto di pagamento a piè di lista del sistema sanitario.

tra le Regioni in funzione del meccanismo di distribuzione del Fondo sanitario (tanto per intenderci la quota *pro* *capite*) e, per un 20 per cento, destinato a quelle Regioni che comunque solo adesso, e in modo retroattivo, procedono a piani di rientro che permettano loro di coprire il disavanzo sanitario. Immagino che questo procedimento sarebbe più equo e solidale, signora Ministro, e non permetterebbe di disperdere al vento il patrimonio di cultura amministrativa che in questi anni,

Signor Presidente, l'emendamento proposto mira ad eliminare la disparità di trattamento che il provvedimento in questione ha creato nei confronti delle Regioni, ma soprattutto nei confronti dei cittadini. dei cittadini. È inaccettabile che si continuino a premiare le Regioni che creano disavanzo a danno di quelle virtuose, come il Veneto, indicato non da Forza Italia ma dall'Organizzazione mondiale della sanità come un esempio da seguire. È singolare che si tolgano finanziamenti e quindi prestazioni a chi opera meglio. Non si nasconda il Ministro dietro un concetto di solidarietà. È falso. E' un provvedimento che favorisce soltanto alcune realtà *(Applausi dal dell'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini e senza prevedere l'attivazione di alcun controllo. Con questo provvedimento si penalizzano i cittadini che in alcune Regioni perderanno servizi essenziali e si avvantaggiano altre Regioni e i loro apparati, come il Lazio e la Campania, senza che vi sia un controllo rigoroso sulla spesa e senza un vantaggio certo e reale in termini di servizi. non si riorganizza il servizio sanitario con provvedimenti a pioggia indiscriminati - così si nega, si blocca lo sviluppo - ma solo responsabilizzando i comportamenti di spesa regionale, come avevamo fatto

ricorrere ad un concetto di responsabilità. È una cultura, quella della responsabilità, che manca - in questo settore come in altri - a questo Governo e che porterà i cittadini ad avere sempre più sfiducia nelle istituzioni per quella scarsa attenzione che oggi le stesse, come questo Governo, hanno nei confronti dei bisogni reali dei cittadini.

che stanno alla base del parere contrario che il Governo intende esprimere sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.505 e di quello governativo 1.0.200. Per opportunità di sintesi, gradirei lasciare una memoria scritta con la quale si dà piena argomentazione delle ragioni che intenderei ora sinteticamente riassumere. L'obiettivo del provvedimento è quello di porre rimedio alla latente crisi finanziaria, senza pregiudicare il conseguimento degli obiettivi per il Patto della salute che sono stati enunciati per l'anno in corso e per gli anni successivi. della crisi finanziaria è tale per cui non è immaginabile poter utilizzare le risorse correnti per ripianare i debiti passati. Allo stesso tempo, preciso intendimento è quello di attuare dei concreti interventi che impediscano la formazione degli squilibri finanziari nel futuro. Le caratteristiche del provvedimento, nella sua integrità, che quindi inducono a non accogliere alcune modifiche emendative che ne cambierebbero l'impianto generale possono essere sinteticamente ricordate nei seguenti punti: innanzitutto, si tratta di una manovra di finanza straordinaria che ripartisce su un arco temporale adeguato, realisticamente adeguato, gli oneri del ripiano dei disavanzi che rimangono a carico delle Regioni. Va ricordato appunto anche l'obbligo di applicare le aliquote massime di prelievo per poter generare risorse finanziarie sufficienti. Il secondo punto - particolarmente qualificante - è che il criterio di riparto è mirato a far accedere al al provvedimento solamente le Regioni per le quali sono in atto le cosiddette procedure di affiancamento; quindi, modificare i criteri di riparto significherebbe estendere anche a Regioni per le quali non è in atto la procedura di affiancamento. La procedura è particolarmente importante perché vengono definite le azioni correttive, non solo finanziarie ma anche riconducibili a quello che può essere definito un piano industriale, e mirate proprio ad evitare che anche nel futuro si costituiscano gli elementi che stanno alla base dello squilibrio finanziario. Quindi, vi è un'azione coercitiva che il Governo impone in capo alle Regioni e che si estrinseca in particolari interventi in funzione delle particolarità e delle cause particolari che sono alla base della generazione dei disavanzi. Quindi accogliere criteri diversi significa di fatto stravolgere completamente l'impianto del provvedimento nella sua interezza; non solo, significa anche

correttive che obbligatoriamente devono essere fatte. Alcuni dei piani sono stati già firmati con le Regioni. Sono già stati sottoposti criteri di riparto alla Conferenza unificata Stato-Regioni, per cui modificare l'impianto del decreto significherebbe vanificare questa accurata azione, sinora intrapresa. Questa è la motivazione che induce il Governo ad esprimere parere contrario non solo a questi emendamenti, ma anche agli altri che verranno successivamente discussi. Mi riservo - ripeto

e in gran parte non può che essere condivisibile, avendo egli enunciato dei princìpi che non possono che essere universali nella politica, soprattutto quando si parla di solidarietà e di privilegiare la qualità;

questo provvedimento sta di fatto premiando proprio i meno meritevoli, quindi sta disincentivando quelle Regioni cui molti di voi che invece autonomamente, avendo sforato la spesa sanitaria, hanno deciso di fare un piano di rientro, con un intervento coraggioso, non solo sulle spese ma anche sull'IRPEF e sull'IRAP. Quindi, quello che stiamo cercando di far capire è che tutta questa grande benevolenza che state ostentando è diretta esclusivamente a quattro Regioni, alle quali state chiedendo un piano di rientro ma senza fissare quei paletti e quelle garanzie che credo siano doverosi nei confronti di Regioni Regioni sfuggite a qualsiasi controllo e che hanno una spesa sanitaria eccessiva, proprio perché sono state incapaci di creare dei controlli. Quindi, non siamo

Anche se nei prossimi emendamenti potrò illustrare ulteriormente il concetto, chiedo che voi votiate favorevolmente questo emendamento, che interviene solo per correggere in senso qualitativo il provvedimento che state portando avanti.

Presidente, la Lega Nord voterà a favore di questo emendamento. Ricordiamo che questo provvedimento costa ai padani e agli italiani più di 50 euro a testa,

in questo provvedimento non paga nessuno, non paga nessun dirigente. Ci sono dirigenti delle ASL assunti per evidenti motivi politici,

che va in un determinato posto al Paese.

Volevo semplicemente sottolineare il fatto che, probabilmente, o il Ministro abita in un altro Paese o non conosce la realtà dei fatti: io non capisco veramente che cosa ci sia di federalista, che cosa ci sia di richiamo alla responsabilità in un provvedimento che semplicemente prende i soldi da una parte del Paese e li regala ad un'altra parte senza un minimo di richiesta di senso di responsabilità. Ricordo che 3 miliardi non sono propriamente una cifretta. Capisco - come ho detto in altre occasioni - che quando si parla dei soldi degli altri chi se ne importa, però 3 miliardi di euro, per intenderci, è quanto costerebbe per esempio la BREBEMI, cioè quell'autostrada che eviterebbe a 300.000 bergamaschi di lontana memoria di passare ogni giorno tre ore al mattino e tre ore alla sera per andare semplicemente a lavorare e pagare le tasse con cui si coprono questi 3 miliardi. Quindi, con un provvedimento che vuol farsi passare sotto silenzio e che va solo a mettere una pezza, a coprire un buco, per esempio, per una Regione che può essere una Regione-Stato come la Lombardia, che aspetta da vent'anni un'autostrada che permetta ai suoi cittadini di lavorare, buttiamo via l'equivalente di quanto basterebbe a fare questa opera pubblica. Allora, signor Ministro,

*(LNP)*. Signor Presidente, lei correttamente, in base a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo di ieri, ha richiamato già due volte - ribadisco: correttamente - il mio Gruppo al rispetto dei tempi. Però qui si sta evidenziando una questione: la *ratio* del contingentamento dei tempi, soprattutto quando siamo in presenza di un decreto-legge, credo sia quella di evitare che l'opposizione, o comunque le parti politiche che non vogliono a nessuno costo far passare un provvedimento,

oppure sono imbarazzati e non sanno come giustificare questo provvedimento che manderà i soldi, come ha dichiarato credo opportunamente il senatore Novi, in parte anche Allora io non credo che la *ratio* del contingentamento sia quella di impedire ai Gruppi di parlare ma, appunto, quella di arrivare ad un voto nei termini stabiliti. Si era stabilito che a questo voto si sarebbe dovuti giungere domani mattina o comunque, nella migliore delle ipotesi, questa sera alle ore 21. Allora io chiedo alla Presidenza di interpretare la decisione dei Capigruppo in questo senso e lasciar parlare chi vuole parlare, e quindi non coartare il dibattito, perché non credo sia questa la *ratio* del Senato, in modo che si voti questa sera alle ore 21. Chiedo che, se qualcuno ha qualcosa da dire, possa farlo senza essere costretto nella camicia di forza di un contingentamento che tra l'altro non vuole, come ho già detto, coartare il dibattito ma semplicemente garantire il voto nei termini previsti.

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale Ciò che si sta dibattendo in quest'Aula è già stato fatto: abbiamo già provato ad intervenire. Io ho con me gli interventi dei deputati del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania - se avrò ancora l'opportunità di intervenire, li espliciterò - che dicono quanto sia inutile

o che si intervenga sull'IRPEF e sull'IRAP o che utilizzeremo i nostri ammalati come un bancomat da prosciugare. Il è questo: di fronte a Regioni che in tutti questi anni, contrariamente ad altre Regioni, non hanno approntato alcun piano di rientro, alcun intervento, noi oggi diamo benevolmente 3 miliardi di euro, senza chiedere minimamente delle garanzie. Sarebbe stato legittimo - e credo sia legittimo chiedervelo - che questo atto fosse contemporaneo alla presentazione di un programma, ad una messa messa in atto di tutti quei provvedimenti che voi auspicate ma che non sono garantiti. Io veramente rimango a bocca aperta perché state dando un assegno in bianco a chi già ha usato assegni a vuoto.

fino a un mese fa aveva certificato il bilancio con un buco di 320 milioni; dopo dieci giorni questo bilancio era di 1 miliardo e 950 milioni di euro. Questi signori non hanno parola: almeno stendiamo nero su bianco la promessa del rientro.

anche solo per il motivo di far presente loro, nella maniera più diretta possibile (cioè costringendoli a mettere mano al portafoglio), ciò che i loro amministratori stanno facendo. In fin dei conti, quegli amministratori non si comportano correttamente perché non rispondono di persona

oltre a misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, nuove compartecipazioni dei cittadini alla spesa sanitaria, non sia altro, al contrario di quanto ci ha detto il Ministro poco fa, che l'unico sistema di responsabilizzazione dei cittadini e quindi delle amministrazioni più vicine ai cittadini stessi - in questo caso le Regioni - per far sì che ci sia un diretto controllo da parte della cittadinanza alla spesa. Quale sistema migliore che quello di legare appunto la spesa sanitaria e il recupero del *deficit* sanitario nelle Regioni ad un incremento fiscale

in maniera corretta, perché è giusta la sottolineatura che da ultimo ha svolto il collega: la solidarietà non può essere disgiunta dalla responsabilità. Il problema, però, è che la compartecipazione ulteriore da parte dei cittadini purtroppo in alcune Regioni italiane si è già determinata,

Allora qual è il problema fondamentale? Premetto che non vorrei che qualcuno all'interno di quest'Aula volesse apparire più responsabile dei solidali senza responsabilità e più solidale dei responsabili senza solidarietà. Prendo atto che, nella memoria storica e nella responsabilità delle forze politiche, c'è anche chi dimentica di aver avuto assessori in quelle Regioni dove si sono determinati gli sfasci di carattere sanitario;

fondamentale è di sanzionare quelle realtà dove tutto questo è frutto di spreco e di mala gestione e distinguere anche quelle situazioni in cui una parte di spesa sanitaria è determinata da criteri di riparto

bisogna tenere conto. Credo che qualcuno debba considerare questo, perché c'è un sistema di riparto iniquo che, insieme allo spreco, che va sanzionato, determina condizioni a cui con equilibrio e responsabilità bisognerebbe tutti guardare.

dichiarazioni fatte in quest'Aula dal Sottosegretario sulla metodologia di attuazione dei piani di rientro, che in base alle considerazioni espresse questi sembrerebbero

è temporalmente sfalsato. Questo è un fatto che ritengo sia necessario mettere in dovuta evidenza in quanto non si possono rappresentare delle procedure come trasparenti quando, in realtà,

Turco) andrebbe a copertura della cosiddetta decurtazione del *ticket* dei 10 euro, aggiungo che la cifra di 811 milioni di euro era stata demandata completamente a carico delle Regioni, che avrebbero dovuto provvedere a coprire queste risorse. Sembra - sottolineo «sembra» - che il Governo abbia intenzione, attraverso uno pseudo-accordo con le Regioni, di coprire questo disavanzo per una cifra equivalente alla metà.

di ricorrere alla suddivisione *pro capite* e non allo stanziamento come stabilito nella procedura presentata dal Governo.

Presidente, nell'emendamento si richiede il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità. Il Patto di stabilità è un atto che dev'essere rispettato universalmente in tutto il Paese da tutti gli enti locali. Votare contro questo emendamento significa creare delle zone di extraterritorialità

che, contrariamente a quanto si pensa, in realtà la sanità non è sostenuta dalle tasse locali nel senso che tutti gli enti locali pagano comunque alla cassa centrale e quest'ultima redistribuisce In questo modo viene a mancare qualsiasi collegamento di responsabilità diretta per cui arriviamo a situazioni come, per esempio, quella del Fondo di solidarietà nazionale, pagato al 57 per cento dalla sola Lombardia, o quella dell'IRAP che dovrebbe sostenere

salsa. Mi sembra che la Conferenza Stato-Regioni sia titolata dalla Costituzione a dover intervenire in materia e chiediamo che la stessa possa almeno essere sentita.

Si è parlato di piani di rientro stabiliti con le Regioni. D'altro canto, ricordiamo che l'accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 prevede un meccanismo al quale lei prima ha fatto riferimento. Del resto, avete reinserito in finanziaria, nel patto per la salute, questo meccanismo che è diventato cogente. Adesso naturalmente ci aspettiamo di verificare come commisurate lo stanziamento destinato ad alcune Regioni e i piani di rientro di queste Regioni con le normative vigenti, cioè l'innalzamento dell'aliquota IRPEF e IRAP a totale copertura del disavanzo. La domanda, e la riflessione che pongo a tutti i colleghi, è se tutti si sono resi conto di cosa significhi questo passaggio perché, nonostante le risorse stanziate da questo eventuale provvedimento siano consistenti, la copertura a totale disavanzo che dovrà essere attuata, sia pure in senso pluriennale, con l'incremento delle quote dell'IRPEF e dell'IRAP, rappresenta per alcune Regioni un elemento di fortissima criticità per quanto riguarda il livello di tassazione. Voglio ricordare che nelle precedenti leggi finanziarie, quelle del Governo Berlusconi (mi riferisco soprattutto all'allora sottosegretario Vegas le seguiva), le Regioni fecero sempre delle battaglie consistenti per quanto riguarda il vincolo di non incremento delle aliquote IRPEF e IRAP. era il seguente: lo Stato centrale riduce la pressione fiscale, le Regioni o gli enti locali non devono invece, in modo surrettizio, sostituirsi a livello di pressione fiscale allo Stato centrale; cosa che onestamente, al di là dello specifico provvedimento,

nell'ambito dell'attuazione di questi piani di rientro, qual è l'aliquota IRPEF e IRAP che le Regioni dovranno inserire per coprire il disavanzo.

come, a differenza di qualsiasi altra suddivisione di risorse finanziarie, nell'ambito del Sistema sanitario nazionale le Regioni abbiano sempre avuto l'opportunità, il modo di discutere e di partecipare alla valutazione di come attribuire le risorse disponibili alle singole Regioni.

destinate sono state definite in funzione dei piani di rientro, cosa che invece avrebbe dovuto avvenire esattamente in modo opposto. Ma questo, l'ho già detto, è una delle tante storture di questo provvedimento. In buona sostanza - torno a ripeterlo

ricordo che stiamo parlando di un provvedimento che mette a disposizione 3 di euro solo per quattro Regioni. Quindi, valutate la possibilità di votare favorevolmente quegli emendamenti che mettono in condizione altre Regioni che hanno gli stessi problemi - vedi la Sicilia e altre - di poter partecipare anch'esse a queste agevolazioni e a queste finalità. Ripeto, questo decreto non può discriminare e, soprattutto, discriminare come adesso, favorendo cioè chi ha sforato di più e non invece quelle Regioni

Presidente, ho appreso in questo momento che si è verificato un ulteriore incidente sul lavoro nella mia cittadina di Grosseto: un Comune di meno 70.000 abitanti che nel giro di quindici giorni ha già visto due morti, uno schiacciato dal carrello di mattoni nella fornace di San Martino poco tempo fa ed oggi nel centro cittadino un altro operaio schiacciato dalla ruspa mentre lavorava alla manutenzione della rete fognaria. È un livello, questo sì, di insicurezza intollerabile che credo impegni tutti noi, le istituzioni ed il Parlamento a dare risposte concrete perché finisca una volta per sempre questo infinito elenco di morti che tutti i giorni insanguinano le nostre strade, molte volte per riuscire solamente a malapena a sostenere una famiglia e a guadagnare un tozzo di pane. *(Generali

Speravo che vi fosse una circostanza diversa per chiedere quello che sto per chiedere, intanto per l'attività costante, quotidiana che svolge la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. A me dispiace che il collega Castelli ne sappia poco; probabilmente una maggiore partecipazione del rappresentante della Lega potrebbe dare elementi e notizie precise su quello che stiamo facendo continuamente. Desidero sollecitare il Governo a rispondere a quanto ha chiesto all'unanimità la Commissione. Il Governo da una mese ha precise richieste, indirizzi da sviluppare e da porre in essere: non abbiamo il piacere di una risposta. che questo sia un fatto non polemico da cogliere, ma una richiesta, perché sembrerebbe altrimenti che questa Commissione non batta un colpo! Ministro Turco, questa Commissione le ha scritto un mese fa: non abbiamo avuto una risposta. Ministro del lavoro, questa Commissione ha scritto un mese fa: non abbiamo avuto una risposta. Lo stesso vale per il presidente del Consiglio Prodi e per il Presidente della Repubblica, cui puntualmente abbiamo indicato percorsi da seguire. Mi auguro che questo fatto solleciti e faccia in modo che non vi siano solamente momenti di dramma e di compianto, ma si agisca!

qui si dice che chi ha avuto....

L'emendamento del Governo è apprezzabile perché supera un momento di difficoltà eccezionale che c'è stato, prende atto di questo fatto e interviene per ridurre i *ticket* per i cittadini, i famosi *ticket* di 10 euro sulle richieste diagnostiche. Quindi, si tratta di un intervento molto importante e apprezzabile del Governo. A questo emendamento del Governo propongo un subemendamento un subemendamento che, credo, vada nella direzione della scelta voluta dal Governo stesso, cioè arrivare all'eliminazione del *ticket* di 10 euro sulle richieste diagnostiche. D'altra parte, vi è continuità con un'iniziativa che 50 senatori del centro‑sinistra hanno assunto qualche settimana fa scrivendo una lettera al Presidente del Consiglio, con la quale si chiedeva

tale impostazione. A me sembrerebbe un errore, giunti a questo punto, con la volontà del Governo che vuole diminuire il *ticket*, lasciare un meccanismo burocratico che, per funzionare, probabilmente costerà di più dell'introito del *ticket* rimanente per le aziende sanitarie locali e per le Regioni. Quindi la mia proposta è un intervento finanziario con questa norma che abolisca completamente il *ticket* senza aspettare il 2008, come il Governo come il Governo annuncia. Vi è un altro rischio che è collegato con tutta la discussione che abbiamo svolto su questo provvedimento. Diverse Regioni, per rientrare dal *deficit,* hanno assunto misure molto forti d'impegno sui loro cittadini ed ora non hanno risorse concrete per abolire definitivamente questo *ticket.* Potremmo quindi trovarci in una situazione di disparità nel nostro Paese

accettare l'abolizione definitiva, con relativo finanziamento, del *ticket* di 10 euro, già da subito, di non aspettare il 2008. Chiedo soprattutto al Senato e all'Assemblea di rispondere positivamente a questa richiesta che è in parte una richiesta del Governo ma è anche una richiesta molto forte dei cittadini italiani.

non intervengo in questa sede sul subemendamento in discussione ma farò delle dichiarazioni quando la Presidenza porrà in votazione l'emendamento del Governo.

Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per avanzare una proposta. Lei, i colleghi e anche il Governo ricorderete che quando sono stati letti i pareri sugli emendamenti è stato annunciato un parere contrario della 5a Commissione sull'emendamento del Governo di cui la proposta del senatore Mazzarello costituisce

ma sotto il profilo qualitativo la soluzione è la stessa. Ora, senza far perdere tempo a lei e all'Assemblea con l'illustrazione delle ragioni tecniche per cui quella copertura ha ricevuto parere contrario, le chiedo di rinviare la votazione su questo emendamento aggiuntivo del Governo, con relativi subemendamenti, alla seduta di oggi pomeriggio perché, nel corso della discussione, pur avendo la Commissione formulato parere contrario senza riferimento all'articolo 81, è stato rivolto un è stato rivolto un invito pressante al Governo a cambiare la formula di copertura. Naturalmente, questo non è ancora avvenuto però vi proporrei di riunire la Commissione bilancio per esaminare un'eventuale proposta Per questa ragione la pregherei, signor Presidente, di rinviare alla seduta di oggi pomeriggio la votazione sull'emendamento del Governo e sui relativi subemendamenti. Non vorrei che facessimo dei pasticci che

Presidente, pur apprezzando le sue qualità e il pragmatismo con cui presiede questa seduta e altre in precedenza, ho da porle un problema.

Signor Presidente, il problema è proprio quello sollevato dal collega Paravia, perché lei ha ragione a dire che è stato votato il testo 2 dell'emendamento 1.505, tuttavia il testo 2, per un accordo intervenuto tra i Gruppi,

Questo era il testo dell'emendamento (sul quale c'era accordo tra maggioranza e opposizione) recepito dal relatore. Si era discusso su una modifica più ampia, ma alla fine si era convenuto che l'unica modifica accessibile fosse rappresentata dal testo 2 dell'emendamento 1.505, con la semplice modifica dell'eliminazione delle parole «o proseguite. ». Questo era ciò che l'Aula sapeva fosse stato messo in votazione. Capisco la concitazione del momento ma, Presidente, è evidente che è necessario il raccordo tra quello che lei formalmente mette in votazione e quello che l'Aula sa che viene messo in votazione. L'Aula, proprio perché soltanto dell'emendamento 1.505 si era discusso a lungo, era perfettamente consapevole che il testo

Senatore Manzione, il Parlamento non vota per tradizione orale, ma vota testi scritti e il testo scritto è quello che è stato votato.

che abbiamo consegnato era esattamente quello posto in votazione (il Senato per sua natura sa sempre ciò che vota, perché - come lei ha detto - vota testi e nel testo non c'era nessuna modifica), è vero che stavamo cercando di ragionare ancora, ma il testo depositato era quello che abbiamo votato: testo sul quale, per la verità, abbiamo discusso molto. Purtroppo, non si è arrivati in Commissione a un voto finale. Quindi, da una parte ribadisco la correttezza formale del voto e il carattere

In sede di coordinamento non si modifica il testo di un emendamento che è stato votato in un determinato modo: non siamo al Consiglio comunale di Canicattì, con tutto il rispetto per il Comune di Canicattì. Quindi, delle due l'una: o si accetta quel tipo di soluzione che non ci trova d'accordo complessivamente sul testo oppure il Governo può presentare quando vuole, e se è d'accordo, un emendamento. Lo può fare oggi pomeriggio e in quella sede noi potremo esprimere il nostro parere.

per dare all'Aula una notizia molto brutta di cui credo il Senato

giudizio, nell'orgia di dichiarazioni sulla famiglia, sui bambini e sui minori che quotidianamente maciniamo, sarebbe un gesto importante ottenere dal Ministro e da questo ramo del Parlamento l'impegno, fra le molte cose ambiziose che declamiamo, a limitare la libera circolazione in questo Paese civile di vere e proprie belve. che nessuno vuole ucciderle, ma è inaccettabile che vengano tenute da privati cittadini che non sono in grado di controllarle, soprattutto quando azzannano e ammazzano i nostri bambini. Oggi a Torino, tra l'altro, è stata azzannata anche la nonna Non è una evasione dalle cose importanti che stiamo decidendo, ma credo che questo sia un fatto di cronaca che deve entrare in quest'Aula e investire la responsabilità del Governo, anche perché si tratta